L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

sabato dalle ore 9 alle ore 14, per poi riprendere lunedì. Signor Presidente, io chiedo il suo autorevole intervento e dichiaro pubblicamente che il mio fisico non regge a questo ritmo, essendo io un parlamentare che le carte le vuole assolutamente leggere. Il problema è un altro: noi chiediamo un accordo, nella dignità delle singole posizioni culturali; se si vuole lo scontro, ci possono anche far tacere e così si arriverà

in Commissione affari costituzionali lo stesso relatore del parere di costituzionalità sul disegno di legge inerente

In sede di Ufficio di Presidenza, presenti i Capigruppo, si è stabilito il calendario per permettere alla Commissione di espletare il suo lavoro, affinché si

una nuova finestra"). Ricordo, come del resto tutti i senatori già sanno, che le Commissioni sono autonome nell'organizzazione dei propri lavori. In ogni caso, mi farò carico di riferire al Presidente le osservazioni che sono state qui espresse dai colleghi senatori.

la convinzione che ci troviamo davanti ad un ennesimo caso emblematico del degrado della qualità della produzione legislativa del nostro Parlamento. Noto che si tratta di un degrado progressivo. Non è una malattia che si manifesta oggi con questo provvedimento, ma è una malattia che viene da lontano e che, negli ultimi tempi, ha assunto un ritmo di aggravamento molto veloce e ormai presenta, dal mio punto di vista, le caratteristiche evidentissime della malattia incurabile ed inarrestabile.

Il Governo dispone in Parlamento di una solida maggioranza che gli consente naturalmente di attuare i suoi programmi e di lavorare in sicurezza politica e parlamentare.

che non può che portare, e infatti fatalmente porta, ad una legislazione di qualità scadente. virgolette, perché purtroppo spesso si tratta di ragioni dense di ipocrisia politica.

il metodo della decretazione utilizzato dal Governo. Con ciò si è arrecato il massimo insulto al Parlamento: i Regolamenti parlamentari sono usati come argomento dal Governo per non andare in Parlamento. Già nel titolo di questo provvedimento vediamo le tracce, le impronte digitali di questo modo di fare e di governare. Stamattina ho ascoltato, con attenzione, il senatore Malan,

il senatore Malan era a disagio mentre elencava le materie che questo provvedimento disciplina o vorrebbe disciplinare. che contiene nel suo titolo «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», signor Presidente, non dovrebbe essere esaminato dal Parlamento

per stratificazioni successive. Infatti, ad un provvedimento sullo sviluppo economico, si è andata progressivamente sommando una messe di argomenti, di normative, un numero elevatissimo di questioni

discussione generale a parlamentari che non hanno la possibilità di conoscere nell'interezza il provvedimento di cui debbono parlare e su cui debbono esprimersi. Signora Presidente,

con titoli sulla semplificazione che contengono deleghe senza alcun limite e senza alcuna definizione precisa dell'oggetto - come costituzionalmente sarebbe necessario - e senza nessuna delimitazione dell'azione del Governo.

lungo tempo a discutere e sulla quale si sono confrontate tesi opposte, ma tutte degne di essere valutate ed esaminate. Noi invece vediamo comparire qui una delega al Governo, anch'essa senza delimitazione e senza definizione. Accanto alle norme sull'ambiente vediamo norme sulla cooperazione internazionale. Poi compare, non si sa perché, signora Presidente, una norma sulla ristrutturazione dell'ENIT e

intervenire in quel provvedimento? Perché, a distanza di poche ore, il Parlamento viene richiamato a discutere la stessa materia in altra sede, con una protesi ad un altro provvedimento? inoltre, norme sulle sedi diplomatiche e consolari, norme sulla tutela dell'utente, sugli sprechi di carta nella pubblica amministrazione,

sterminata. Anche questa delega non ha nessuno di quei paletti che la Costituzione impone ai provvedimenti delegati.

e invece noi viviamo in Parlamento stretti in una morsa tra 39 decreti-legge, voti di fiducia e maxiemendamenti e adesso ripetiamo, per l'ennesima volta, deleghe ampie, sterminate, senza paletti e senza confini. Ma che tipo di legislazione vogliamo fare? Ma come possiamo pensare di dare ai cittadini italiani delle leggi comprensibili,

a macchia di leopardo, di alcune parti del codice di procedura civile. Sino a ieri, in Commissione giustizia, il Ministro della giustizia ha rivendicato

che funzioni e che sia in grado di dare risposte ai cittadini e agli imprenditori in tempi celeri e certi. Una giustizia che ritarda la sua risposta ed è

Ritengo che questa mattina il senatore Berselli, presidente della Commissione giustizia, abbia voluto farci una simpatica provocazione: per

tre disegni di legge organici di riforma della procedura civile non facevano altro che utilizzare il proficuo lavoro svolto, nella scorsa legislatura, in Commissione giustizia del Senato, che era pervenuto, con un accordo condiviso di tutte le componenti politiche, ad un testo frutto di un lavoro estremamente completo.

tecniche e tattiche dilatorie, è esattamente il contrario: noi nella riforma della procedura civile non solo ci crediamo, ma la vogliamo; voi volete invece fare una cosa diversa. Penso che per la prima volta nella storia del Parlamento la riforma della procedura civile sia stata esaminata, alla Camera, dalla Commissione giustizia in sede consultiva provvedimento era assegnato alla Commissione bilancio; credo sia la prima volta nella storia del Parlamento italiano che una riforma di sistema

peraltro, ne sono stati annunciati altri, che ancora non conosciamo, da parte dei relatori. Questo lungo parto di riforma della procedura civile

a decreti legislativi da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Quale urgenza per assicurare lo sviluppo del Paese! Non avete fatto una riforma:

dai disegni di legge organici che noi avevamo presentato e l'avete prospettato come riforma. Sono furti continui delle idee altrui, disseminati tanto per fare qualche cosa. No, la vostra non è una riforma, la vostra non è una riforma, è soltanto un intervento con ritocchi disaggregati, senza una visione complessiva che riguardi veramente la riforma del processo civile. Anche se alcuni aspetti, essendo rubacchiati, si ritrovano negli altri disegni di legge, manca una visione d'insieme, manca una visione strategica di ciò che si vuol fare. evidentemente avete dimenticato - il senatore Berselli in questo ha pessima memoria - che dal 2001 al 2006 della giustizia civile non vi è importato nulla, nulla, così come della giustizia penale. Avete soltanto fatto leggi *ad* *personam*, poi accusate noi per aver governato un anno e mezzo e prodotto una serie di interventi normativi non andati a compimento per la fine della legislatura. Volevamo ripartire da lì. Voi volete continuare a spendere degli *spot* ma non avete a cuore la vera riforma della giustizia e quindi non avete a cuore l'interesse dei cittadini. Preannuncio che il nostro voto sarà totalmente contrario.

mi rendo perfettamente conto - ancor più dopo aver ascoltato gli interventi del senatore Zanda e del senatore Li Gotti e del senatore Li Gotti - di come un provvedimento che rechi disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività del Paese, Paese, nel cui impianto vengano innestate modifiche inerenti la materia del processo civile, possa sollevare perplessità in quest'Aula. D'altro canto, lo scetticismo e un certo spaesamento sono comprensibili; sono comprensibili nei colleghi che faticano a confrontarsi con il virtuoso pragmatismo, costume di questa maggioranza. Nonabbiamo dimenticato come alla prova dei fatti ad autorevoli esponenti della parte politica oggi all'opposizione persino la raccolta dei rifiuti urbani apparve un'emergenza inestricabile, sicché un capoluogo di Regione venne umiliato, degradato all'oscena condizione di immondezzaio a cielo aperto. In qualche settimana, onorando la virtù del fare a cui poc'anzi mi riferivo, il Governo, sostenuto da questa maggioranza, cancellò la iattura ripulendo la città. Nonesco dal tema, colleghi senatori. Riaprire un capitolo vergognoso e doloroso di inettitudine e di malcostume non allontana dall'argomento che stiamo trattando, perché la filosofia che sottende l'azione di Governo anche riguardo al decreto-legge n. 112 del 2008 resta quella di mirare al risultato, mentre altrove qualcuno si sofferma su aspetti accessori. Non c'è che dire, sarebbe formalmente più elegante comporre per ogni materia riforme articolate e generali, e questa maggioranza è comunque l'artefice di cambiamenti mai neppure adombrati dal dopoguerra ad oggi; tuttavia, ad un ordinamento complesso e arcaico qual è il nostro, si addicono anche interventi parziali ma efficaci, per per quanto apparentemente estemporanei o persino un po' forzati, *opportun**e et importune*, a tempo e controtempo, per usare un'espressione dell'Apostolo delle genti. Non ci scandalizzeremmo, d'altro canto, neppure se l'Atto n. 1082 non giacesse in Senato da ottobre e se dunque non fossero stati così ampi i tempi per apportare le variazioni del caso alle disposizioni sul processo civile. Se scandalo esiste, infatti, è tutto relativo a ben altra tempistica: come non pensare ai quasi 3.200 giorni mediamente necessari nel Belpaese per portare un processo a sentenza? Una cadenza funebre, in ulteriore e progressiva dilazione. Inoltre, è palese, pienamente avvertito da tutti i cittadini, lo stato di necessità che ha indotto il Governo a intervenire nello spirito di concretezza evidenziato da altre circostanze come quella esemplare a cui ho voluto prima riferirmi. Ci troviamo in un'urgenza obiettiva e talmente sentita che anche l'Associazione nazionale magistrati, non particolarmente tenera con il centrodestra, ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva su questo provvedimento, pur esortando il legislatore ad incamminarsi con maggior decisione sulla strada intrapresa della velocizzazione dei processi. La *ratio* che sottende tali disposizioni, cioè la semplificazione ed accelerazione delle procedure (questo si legge nella nota della giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati), è certamente condivisibile. Ancora in tale nota si afferma che la previsione contenuta nell'articolo 50, a proposito della cancellazione ed estinzione della causa civile dal ruolo, è senz'altro condivisibile poiché consente al giudice di estinguere d'ufficio processi rinviati e cancellati per assenza delle parti, impedendo in tal modo il mantenimento di pendenze fittizie a fronte di una concreta carenza Si aggiunge che anche le novità introdotte dall'articolo 53 in tema di razionalizzazione del processo del lavoro devono essere viste con favore. Questo dice l'Associazione nazionale magistrati. Quanto all'articolo 51, che introduce nel processo civile l'informatizzazione delle comunicazioni e notificazioni alle parti ed ai consulenti, la medesima Associazione non ha difficoltà a riconoscere che si tratta di di una riforma da sempre auspicata dall'Associazione stessa, che consentirà agli ufficiali giudiziari di gestire il carico sempre più gravoso di adempimenti che determinano ritardi nella trattazione dei processi per difetti di notifiche. Non voglio, peraltro, nascondere come il giudizio complessivo di questa associazione di categoria sulle disposizioni introdotte sia di parziale soddisfazione: infatti la nota auspica, altresì, un complessivo ed organico disegno di legge in materia. A questo proposito, vorrei rilevare però come, in un certo senso, l'organicità del provvedimento non sia esclusa, ma appaia in un contesto che fa riferimento ancor più alle esigenze del cittadino che a quelle dell'addetto ai lavori; ed è significativo, in quest'ottica, che lo snellimento delle procedure rientri nel pacchetto di misure sulla competitività. Il disegno di legge n. 1082 non è il semplice contenitore *omnibus* che raccoglie di tutto e di più tra quanto serve a porre in essere interventi utili, ma disparati. In realtà esiste una coerenza di fondo in questo disegno di legge che parte dal concetto di sviluppo del territorio. È guardando ad annose necessità delle comunità locali che è stato possibile - persino opportuno veicolare in un unico strumento lo sveltimento del processo civile e la razionalizzazione della burocrazia nelle amministrazioni comunali, l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate e lo snellimento delle procedure per ottenere le autorizzazioni per le medie e grandi opere, la diffusione delle buone prassi nel settore pubblico e la trasparenza delle retribuzioni dirigenziali; e mi fermo qui, ma vi sarebbero tantissimi altri argomenti. concludendo, signora Presidente, si tratta di una costellazione di provvedimenti che gravita intorno ad un nucleo fondamentale: la comunità e il territorio. Con questo disegno di legge, dal punto di vista pratico, si parte dal cittadino, sempre in ossequio al pragmatismo coerente su cui ho avuto modo di soffermarmi, e si approda all'ambito sociale, che richiede un intervento. Di fatto, viene a configurarsi un modo diverso, meno settoriale, per nulla corporativo e del tutto anticlientelare, di indirizzare l'attività di normazione. Nel rispetto di questi valori, colleghi

però, che a questo punto integrerei meglio queste eterogeneità e frammentarietà, già sufficientemente illustrate, mettendo invece l'Aula di fronte allo scandalo del modo in cui questo provvedimento ha marciato:

estratti dal disegno di legge n. 1441, deliberato dalla Camera nella seduta del 5 agosto 2008. Viene approvato dalla Camera come disegno di legge n. 1441-*bis* il 2 ottobre, trasmesso al Senato in data 6 ottobre e assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia in sede referente il 7 ottobre. L'esame in Commissione è, in realtà, iniziato il 15 ottobre 2008, mentre il 4 novembre è stata respinta la richiesta di stralciare gli articoli riguardanti il processo civile, su cui vi ha già intrattenuto il collega Li Gotti. degli emendamenti nelle Commissioni riunite è stato fissato al 19 novembre 2008: si trattava di una scadenza importante, perché il Regolamento del Senato vieta di presentare in Assemblea emendamenti che non siano stati preventivamente depositati in Commissione e respinti. Il relatore e il Governo, dopo questa data, hanno continuato a presentare nuovi emendamenti pressoché ad ogni seduta, fatta salva la facoltà di subemendare accordata ai Gruppi. Nel corso delle sedute dell'ultima settimana, siamo andati avanti nell'esame degli articoli e degli emendamenti, ma vi è stato l'accantonamento di numerosi articoli, nonché la presentazione di ulteriori nuovi emendamenti sia da parte del relatore che del Governo, oltre alla riformulazione di altri già presentati. La Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato il provvedimento in Assemblea quando le Commissioni non ne avevano ancora terminato l'esame

Questo termine, fissato per martedì 24 febbraio 2009, alle ore 17, era infatti riferito solo agli articoli da 1 a 26; quello per gli emendamenti relativi agli articoli da 26 a 45 ci è stato detto che sarebbe stato comunicato successivamente. Mi rendo conto che

cui riferire gli emendamenti, recante alcune modifiche rispetto a quello precedente e soprattutto contenente alcuni significativi articoli aggiuntivi all'articolo 26: si parla di riforma del processo amministrativo, di norme riguardanti l'Avvocatura dello Stato, la Corte dei conti e così via. La Corte dei conti sembra il fantasma che ritorna e attraversa le varie leggi, entrando e uscendo da porte e finestre e rimescolandosi nelle materie. Per emendare tutta questa materia rimanevano pochissime ore, dal momento che il termine delle ore 17 rimaneva invariato. tratta di un vizio che ritorna: abbiamo di fronte dei testi e abbiamo pochissimo tempo, non dico per emendarli, ma anche per leggerli; infatti, per emendare un testo, bisognerà pure avere il tempo di leggerlo e di studiarlo. In seguito alla scadenza del termine, sempre nel pomeriggio di martedì 24, è arrivata la comunicazione ai Gruppi che le Commissioni 1a e 2a avevano terminato l'esame del disegno di legge con altri nuovi emendamenti e riformulazioni del relatore. Allora, è stata data informazione dalla Segreteria dell'Assemblea che finalmente sarebbe stato trasmesso anche il testo degli articoli rimanenti dal 26 al termine, come modificati dalle Commissioni. Nello stesso tempo, si informava che veniva fissato alle ore 19 del 25 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti riferito al totale degli articoli. Nella mattinata di oggi (alle ore 9,10), è stato consegnato il testo finale delle modifiche apportate dalle Commissioni. Questo testo comprendeva anche modifiche ed articoli che precedevano l'articolo 27, nonché tutte le modifiche degli articoli dal 27 al 45. Alle ore 13,30 è stato inviato un fax con correzioni al testo finale e, in particolare, con differenze riguardanti gli articoli 27 e 39. Nell'articolo 39 risultavano inseriti emendamenti che il resoconto di Commissione dava erroneamente per bocciati, mentre non lo erano; tale resoconto è stato quindi corretto *on**line* e gli emendamenti approvati sono stati inseriti nel testo consegnato ai Gruppi,

Poiché si tratta di un esito che, a termini di Regolamento, determina la proponibilità o meno dell'emendamento, si comprende che tipo di confusione questo modo di procedere possa ingenerare nei soggetti, cioè noi che siamo costretti ad occuparci della questione. Se mi permette, signora Presidente, dopo questa inverosimile sequenza di fatti e misfatti, di procedura e di

nasce da un emendamento improponibile per estraneità alla materia e proroga una delega a termine già scaduta; tutto ciò si basa su una potestà opaca del Governo sull'ambiente e il Senato può esprimere solo un parere non vincolante. Qui c'è, *in* *nuce*, un vizio di natura costituzionale: fino al 2011, in virtù di una delega del 2004, vi sarà la procrastinazione ed il rinnovamento della delega, che coprirà ben tre legislature, di un provvedimento del quale in realtà non si conosce la struttura interna.

Signora Presidente, abbiamo sentito dei giudizi aspri, drastici.

fa parte della dialettica, è il gioco delle parti. Tuttavia io amo anche essere onesto e riconoscere a Cesare quel che è di Cesare. Del vero c'è nelle loro lagnanze: si poteva, come si può sempre, affrontare la materia in modo diverso, sicuramente più organico, come effettivamente si dovrebbe affrontare una riforma;

Oggi forse il più importante quotidiano nazionale riporta addirittura due pagine sulla funzione dei magistrati onorari,

Il loro peso complessivo, tra magistrati togati e onorari, è quasi parificato: sono 9.000 i primi e circa 8.000 i secondi, dei quali circa 4.000 sono i giudici di pace.

affiancata a quella togata, sta assumendo un peso importantissimo e a questa oggi noi dobbiamo dare una risposta. I vice procuratori onorari svolgono

oppure alle strutture esistenti, ai consigli degli ordini degli avvocati, mentre gli avvocati stessi avranno l'obbligo di informare i propri clienti della possibilità di adire vie diverse da quelle ordinarie.

su un altro piano rispetto all'utente che deve soltanto accettare condizioni su modulistiche preconfezionate. Infatti, concordando, i Ministeri dell'economia, della pubblica amministrazione e degli affari regionali

Tornando alla magistratura onoraria,

interventi di cooperazione finalizzati al superamento di criticità di natura umanitaria, sociale o economica. Noi continueremo a dare aiuti umanitari e ad operare nella cooperazione allo sviluppo internazionale, però chiediamo un po' di corresponsabilità:

la gestione dei flussi migratori, e sappiamo quanta materia viene trattata in quest'Aula; il secondo annoso problema, che ciclicamente ci ritroviamo, è l'affollamento carcerario. Daremo una mano a quei Paesi che aiuteranno l'Italia in questi due importanti settori. Vorrei ricordare a tutti colleghi della sinistra, che hanno un po' inveito su tali modalità operative, un grande uomo della sinistra, che ricordava al Parlamento che tipo di giudizio andrebbe dato su un Governo:

che, in verità, il presidente Berselli, anche abilmente, ha cercato di ribaltare, dando l'impressione che da parte del centrosinistra vi sia o vi fosse l'intenzione

«Disposizioni per la riforma del processo civile» (Atto Senato n. 1016) in data 15 settembre 2008 e, se qualcuno volesse esaminare questo disegno di legge, vi troverebbe i principi della lealtà processuale, il calendario del processo, l'alleggerimento delle questioni di competenza, il procedimento sommario, la semplificazione del regime delle nullità processuali, l'unificazione dei riti. non solo non siamo affatto indifferenti alla riforma del processo civile, ma dal 15 settembre abbiamo presentato un articolato completo, composto di tutte le questioni che poi, via via, sono state affrontate

a noi pare non condivisibile è inserire un progetto di riforma del codice di procedura civile in un provvedimento legislativo così vasto, eccentrico e lontano dalle questioni che attengono alla giustizia civile.

sulle questioni che attengono all'energia anche per i diritti soggettivi. Vi è quindi una reiterazione nell'errore. Pareva e parrebbe a noi, invece, che tutte queste questioni andassero affrontate in sede referente in Commissione giustizia, nell'ambito di un confronto organico e sistematico, condiviso tra centrodestra e centrosinistra. Oggi, non avremmo un articolo di legge che delega il Governo a produrre mesi norme in materia di unificazione dei riti: forse, da settembre ad oggi, avremmo un elaborato che unifica i riti. Quindi è esattamente il contrario di quanto si è sostenuto. Certo, a giugno è stato facile dire «abbiamo modificato il processo civile»,

esempio, il filtro che riguardava la cosiddetta doppia conforme; è stato inserito il calendario del processo, contenuto anche nel nostro disegno di legge e che avevamo annunciato; si interviene sulla questione della competenza della giurisdizione in maniera efficace, con l'articolo 38 che l'eccezione di incompetenza vada eccepita nella comparsa di risposta depositata e quindi prevedendo un blocco a tutta una serie di questioni intermedie che riguardano il processo.

persa. Possono essercene certo delle altre, però dispiace che su un provvedimento così generale le questioni della giustizia, sulle quali avevamo grande possibilità di condividere il lavoro da svolgere insieme, sia stata in maniera

non la nostra disapprovazione, ma comunque una posizione che da un certo punto di vista, per quanto riguarda il merito, è anche di condivisione, ma si perde in un provvedimento generale che nulla ha a che fare con la riforma della procedura civile.

Onorevole Presidente, debbo dare atto al senatore Galperti di essere stato obiettivo, sereno e anche propositivo. Ascoltando il senatore Li Gotti sembrava veramente che fossimo Alice nel paese delle meraviglie. Il collega Galperti ci ha fatto tornare sulla terra e ha detto che obiettivamente vi è stato un confronto sereno, costruttivo nelle Commissioni riunite e ha dato altresì atto alle stesse Commissioni riunite di aver modificato, migliorandolo, il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Quindi è un confronto, come deve esserci, in un Parlamento democratico, in cui la maggioranza non deve far pesare i propri numeri per soffocare e umiliare l'opposizione. Tant'è che alcuni emendamenti importanti, come quello del calendario, sono stati approvati e sono frutto di un contributo dell'opposizione. Altri passaggi non irrilevanti che abbiamo affrontato in sede di Commissioni riunite hanno portato a modifiche suggeriteci dalle stesse opposizioni. non abbiamo imposto a scatola chiusa un testo blindato tant'è che è stata la stessa maggioranza che ha proposto vari emendamenti al Governo ottenendo dallo stesso una grande disponibilità all'ascolto. Il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - lo sappiamo - non fu esaminato in sede di Commissione giustizia della Camera ma sottoposto soltanto ad un parere. Questa volta la situazione è cambiata, anche in funzione del nostro Regolamento, e abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con il Governo, in particolar modo con il sottosegretario, senatrice Alberti Casellati (che ringrazio per la disponibilità e la partecipazione a tutte le nostre riunioni), con un totale ascolto circa le nostre proposte, a dimostrazione che il testo non era blindato, che non è stato imposto né all'opposizione né alla stessa maggioranza. Non voglio dilungarmi sul contenuto di questo provvedimento, anche perché il relatore, senatore Delogu, ha già sviluppato questo ragionamento nella mattinata odierna. Desidero soltanto soffermarmi su quei passaggi che abbiamo modificato in Commissione, con il consenso dello stesso Governo. Si tratta di aspetti di grande importanza,

prevedeva che non si potesse ricorrere per Cassazione contro la sentenza emessa in secondo grado che aveva confermato quella di primo grado, con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio. In sostanza, laddove vi fosse stata una sentenza immotivata o con una motivazione contraddittoria emessa in primo grado e poi confermata in appello, contro quella sentenza in appello non si sarebbe potuto ricorrere per Cassazione.

brevemente su questo benedetto filtro. Dico "benedetto" perché obiettivamente è stato introdotto in modo assolutamente condivisibile dalla Camera dei deputati, poiché serve per deflazionare il carico di lavoro presso la Suprema corte di cassazione.

sicuramente meglio un unico filtro, rispetto a tanti filtri assegnati alle varie sezioni, per evitare possibili discordanze circa l'ammissibilità o meno dei ricorsi, che potrebbero determinare situazioni davvero imbarazzanti dal punto di vista giuridico. Un altro passaggio che voglio ricordare brevemente, ma sul quale

esso si prevedono due ipotesi. Laddove c'è l'accordo delle parti, c'è la possibilità di chiedere al testimone di far pervenire per iscritto, nel termine fissato, le proprie dichiarazioni.

la richiesta di una sola di esse. La seconda ipotesi che abbiamo previsto è che non vi sia l'accordo delle parti, ma ci sia comunque il controllo del magistrato, a seguito della deposizione, quando si parla di documentazioni di spesa,

Questo era un passaggio molto importante perché abbiamo chiarito la natura di questa testimonianza scritta, abbiamo eliminato gli inconvenienti che avrebbero potuto sorgere in funzione del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e abbiamo dato un contributo positivo e importante

e che noi abbiamo confermato nella sua totalità (eccezion fatta per quella doppia conforme introdotta in Aula alla Camera dei deputati). Il punto è quello relativo alla semplificazione e alla riduzione dei riti.

Noi abbiamo ottenuto dal Governo - e gliene siamo grati - la disponibilità a intervenire in modo pesante per la semplificazione e la riduzione dei riti. quindi ottenuto molto e pensiamo di avere confezionato, insieme all'opposizione e al Governo, un testo ampiamente condivisibile e riformatore.

Ringrazio comunque l'opposizione per la collaborazione e ringrazio i due relatori, i senatori Malan e Delogu, per l'impegno profuso in tutto questo periodo. Ovviamente, ringrazio anche il presidente Vizzini per avere, insieme ai componenti della 2a Commissione, seguito l'*iter* complessivo di un procedimento particolarmente complicato e difficile all'esito del quale siamo consapevoli e orgogliosi di avere presentato un'ottima riforma.

Il senatore Zanda ha parlato di degrado dell'attività legislativa a proposito di questo provvedimento. Noi sappiamo che sicuramente vi è stata un'evoluzione nel modo di fare le leggi

che questi siano positivi, non mi porta a vedere in ciò alcunché di male. Non sono solo le grandi riforme, quelle articolate in tanti bei capi, articoli e titoli,

alcuni - tanti - interventi che vanno a risolvere dei problemi specifici. Credo sia stato svolto un lavoro molto positivo in questo senso,

il nostro settore produttivo e la nostra pubblica amministrazione hanno davvero grande bisogno, specialmente in tempi di crisi economica.

un buono lavoro. Il senatore Divina ha citato, in particolare, le priorità date agli interventi in materia di cooperazione internazionale:

Non c'è nulla di definitivo e di fermo. Se non avessimo portato emendamenti, se non avessimo accettato e votato circa una decina di proposte dell'opposizione ci avrebberodetto

dobbiamo rinnovare il codice di procedura civile, procediamo tutti insieme. Noi siamo pronti a farlo, ma non a sentirci dire che, se portiamo emendamenti, siamo incerti o che, se non li portiamo, blindiamo i provvedimenti. Ritengo pertanto che il testo

Signor Presidente, signori senatori, il disegno di legge che stiamo esaminando - è a tutti noto - origina dall'Atto Camera n. 1441, presentato dal Governo il 2 luglio 2008 alla Camera. Un triplice stralcio operato poco prima dell'aggiornamento estivo dei lavori parlamentari ha generato, tra gli altri, il disegno di legge n. 1441-*bis,* intitolato, tra l'altro, al processo civile, ma in un contesto il cui *incipit* era e rimane: disposizioni per lo sviluppo economico. Non si tratta di un approccio volto a utilizzare la tecnica del provvedimento contenitore, né del prodotto normativo *omnibus,* come questa mattina ha affermato il senatore Casson. Si tratta della consapevolezza, non certo solo del Governo, ma ben diffusa tra tutti i cittadini, del fatto che il lavoro, l'imprenditoria, la libera iniziativa, ma più in generale i rapporti economici e sociali, perfino i rapporti familiari si possono svolgere serenamente e dare i loro pieni frutti in termini di benessere, ricchezza e sviluppo se sullo sfondo l'apparato giudiziario, non solo non dà le necessarie garanzie di tutela rispetto al danno, Voglio citare due fonti, al di sopra di ogni parte, che autorevolmente dimostrano la validità di un approccio che sposa riforma del processo civile e provvedimenti di sviluppo economico. La prima è il rapporto della Banca mondiale del 2007, entrato purtroppo agli onori della cronaca perché è stato impietosamente ricordato che l'Italia è oltre il centocinquantesimo posto nella graduatoria mondiale di efficienza nel giudizio civile, perfino dopo l'Angola e il Gabon. Per la verità, questa posizione tiene conto anche del costo del processo, che in Italia è bassissimo, perché se si guardasse solo alla durata del processo la posizione in classifica scenderebbe ancora. Voglio citare un'altra parte meno nota, ma non per ciò meno significativa, di quel rapporto, quella dove si evidenzia come nei Paesi con adeguate strutture giudiziarie capaci di rendere esigibili i crediti, i fidi bancari crescono del 27 sulla necessità di un sistema giudiziario efficiente, in nome della civiltà giuridica, un sistema che dispensi certezza giuridica agli operatori conviene perché promuove lo sviluppo e il benessere economico. Una giustizia civile veloce fa girare velocemente l'economia. Non sarà un caso - ed è il secondo contributo che volevo ricordare - se la Banca d'Italia, che certamente non ha dirette competenze in materia giudiziaria, ha pubblicato un'interessante ricerca sulle cause di non funzionamento delle riforme del processo civile in Italia con particolare riferimento ai gradi di giudizio successivi al primo. Il nostro istituto centrale è dunque attento alla parte forse più significativa, quella della tutela, del contesto giuridico in cui si muovono i rapporti economici ed esamina diagnosi e terapie che confortano in gran parte l'approccio del Governo. Oggi, il quadro che si presenta è tale che, nella deprecabile eventualità di un qualsivoglia profilo di lite e contrasto tra privati, ciò che lo Stato appresta non è una sede di risoluzione rapida, non è una sede di risoluzione attenta, ma è il vero e proprio inizio di un calvario dove la complicazione prevale sulla complessità e dove costi e tempi si moltiplicano di tanto in quanto si riducono prima le certezze e poi le speranze. Questo è il comune sentire dei cittadini, questo è indegno per un Paese civile. Non si può stare a guardare; il tempo dell'analisi, che è stata ampia e partecipata, ormai è scaduto. Il richiamo del Governo all'urgenza

Il testo pervenuto in Senato è stato esaminato alla Camera dei deputati dalla I e dalla V Commissione. L'esame referente si è svolto durante tutto il mese di settembre fino al dibattito in Aula che si è concluso con l'approvazione il 2 ottobre. È seguita una lunga pausa di riflessione, durante la quale il risultato del lavoro svolto è rimasto all'attenzione di una vasta platea della politica e degli operatori del diritto. A seguito di questa protratta ed intensa attenzione, l'impianto del provvedimento è rimasto intatto nel suo complesso e nelle sue parti principali. In più di un'occasione, inoltre, è emerso l'apprezzamento per un intervento riformatore che era ed è giudicato improcrastinabile e necessario, sia pure con tutti gli indubbi distinguo su taluni aspetti nel merito di singoli istituti. Così mi pare di poter leggere nel parere del Consiglio superiore della magistratura e nell'intervento dell'Associazione nazionale magistrati sui profili della riforma, che vengono giudicati in gran parte condivisibili e certamente, per taluni aspetti, discutibili. Nel complesso dell'esame parlamentare, dunque, l'apporto è stato articolato. Gran parte degli studi del processo civile, elaborati nella precedente legislatura, sono stati trasfusi nell'attuale testo normativo e questo non può essere sfuggito all'attenzione del senatore Li Gotti, perché lo ha ammesso lo stesso senatore Galperti, elencando un numero consistente di istituti presenti nei loro disegni di legge e nel disegno di legge governativo. Il clima ha inoltre conosciuto momenti di sinergia e momenti di approfondimento costruttivo. Di tutto ciò non c'è che da congratularsi con il Parlamento tutto e, per quanto riguarda in particolare il Senato, con i relatori Malan e Delogu, con i presidenti Vizzini e Berselli ed i senatori tutti, sia di maggioranza che di opposizione, cosa che faccio in modo convinto a nome del Governo. Il provvedimento intende dunque perseguire un sistema giudiziario all'altezza di un sistema di sviluppo economico. Obiettivo principale è la riduzione dei tempi del processo civile. È questo obiettivo che costituisce il comune denominatore dell'impianto normativo. Non è una visione strategica, senatore Li Gotti, chiediamolo agli italiani che attendono una risposta di giustizia per 8 o 10 anni. Ho ricordato prima il clamore suscitato dai dati che collocano l'Italia dietro alcuni Paesi africani. Sono altri, per la verità, i dati che mi preoccupano di più: non i raffronti dell'Italia con l'estero, che sono impietosi anche quando sono condotti nell'ambito del più limitato contesto europeo; ciò che veramente preoccupa sono invece i raffronti dei dati italiani nel tempo perché dimostrano che stiamo precipitando nel baratro. La durata effettiva dei primi due gradi di giudizio passa da 2343 giorni nel 1992 a 2565 giorni nel 2001, ultimo anno per cui questi dati sono disponibili.

Rispetto a questo quadro desolante non si può non onorare il senso di responsabilità e realizzare un intervento, perfettibile ed opinabile finché si vuole, come ha sottolineato il senatore Delogu, ma nondimeno necessario in una situazione disastrosa di cui tutto si può dire tranne che può essere lasciata così com'è. La sostanza dispositiva delle norme sul processo civile, finalizzate soprattutto a deflazionare il terribile carico di arretrato che grava su ogni tentativo di scossa del sistema giudiziario, sono ormai note ai senatori ed illustrate nella relazione. Ci sono provvedimenti dal lato della domanda di giustizia, penso in particolare al principio di lealtà processuale, e soprattutto dal lato dell'offerta; un impianto vasto ed articolato che comprende, tra l'altro, le iniziative volte all'unificazione e riduzione dei diversi riti (credo, senatore Berselli, che siano circa una trentina), le norme volte a ridurre i tempi processuali, il nuovo procedimento sommario di cognizione e la mediazione civile commerciale finalizzata alla conciliazione stragiudiziale. Sui giudici di pace, il cui lavoro è da tutti apprezzato, senatore Divina, faremo assieme una riflessione. Qualcosa consentitemi di dire in particolare sul cosiddetto filtro in Cassazione: si tratta di un'innovazione sostanziale e significativa, certo non da tutti condivisa, ma che pare obiettivamente ragionevole, cauta e circostanziata. Ho citato all'inizio un recente studio della Banca d'Italia sul processo civile: ebbene, quello studio, basato sulla letteratura economica, segnala che la complessiva qualità del sistema delle impugnazioni dipende soprattutto dall'efficienza dell'ultimo grado di giudizio, poiché questo condiziona le scelte delle parti e il comportamento dei giudici nei precedenti gradi. In Italia, dice questo studio, i carichi della Corte nel settore civile sono andati aumentando in modo vertiginoso nell'ultimo decennio, mentre le riforme del processo civile hanno,

n. 112, che tra l'altro spingono verso il processo telematico: aumento della velocità, diminuzione dei costi. In cima alla classifica di efficienza processuale, sempre lo studio della Banca mondiale pone i sistemi giudiziari in cui le cause civili possono essere introdotte e proseguite per via informatica. In quei sistemi, si legge nel rapporto, il difensore verifica sul proprio computer il tempo che manca all'udienza fissata e un messaggio automatico sul cellulare lo avverte della convocazione del giudice. In quel tipo di sistema, ci vogliono 150 giorni per definire una causa; nel nostro, 1210: quasi dieci volte tanto. La giustizia civile italiana deve essere portata a livelli di efficienza degni di un grande Paese industrializzato, specie in un contesto generale dove l'ampiezza e la portata della crisi richiedono risposte veloci ed efficaci, capaci nel loro complesso di rafforzare le condizioni di operatività dell'economia. Gli interventi predisposti sono provvedimenti - se si vuole - chirurgici, ma di primo intervento e, soprattutto, mirati selettivamente a ridare mobilità e respiro ad un sistema gravemente compromesso, che non si può assolutamente so che questa consapevolezza è comune - lasciare in queste condizioni. Per questo motivo, auspico l'approvazione convinta di questo progetto. apre una nuova finestra"). È presente in tribuna una delegazione di membri del Congresso della Repubblica del Perù, presieduta dal secondo vice presidente Alvaro Gonzalo Gutiérrez Cueva.